il 12 novembre di quattro anni fa morivano per mano assassina a Nasiriya 19 nostri connazionali. Nella ricorrenza di questo tragico anniversario sono certo di interpretare il pensiero di tutta l'Assemblea aprendo i lavori con un momento di raccoglimento dedicato a quei valorosi figli dell'Italia ed al loro sacrificio. Quella terribile strage lasciò sgomento il Paese, scrivendo una delle pagine più drammatiche, accomunandolo in un dolore intenso e sincero. Oggi, come allora, un'intera comunità nazionale si sente vicina ai loro familiari e rinnova ad essi il sentimento di vicinanza e di affetto mai sopito. L'Italia non ha dimenticato e non dimenticherà mai i martiri di Nasiriya. Non ha dimenticato e non dimenticherà la generosa azione, nella martoriata terra irachena, affinché per quel popolo potesse avvicinarsi una prospettiva di pace, di serena e proficua convivenza, così come l'Italia è unita e si stringe attorno alle donne e agli uomini che, mandati dal nostro Paese nei luoghi dove le guerre ed i conflitti hanno portato morte e distruzione, lavorano con coraggio ed abnegazione perché queste situazioni di dolore e d'ingiustizia scompaiano. Il Senato della Repubblica ricorda oggi con commozione e riconoscenza i caduti di Nasiriya. Invito i colleghi Colleghi, è con dolore profondo che ci associamo al cordoglio per la scomparsa tragica di Gabriele Sandri, un giovane di 28 anni la cui esistenza breve è stata così drammaticamente interrotta. Su questo grave episodio occorrerà stabilire, con chiarezza, colpe e responsabilità e sono certo che ciò sarà fatto con la prontezza e la serietà che una vicenda così drammatica richiede. Un fatto così doloroso non può tuttavia essere, in alcun modo, pretesto per le violenze compiute nella giornata di ieri negli stadi e nelle strade delle nostre città; aggressioni alle Forze dell'ordine, devastazioni, veri e propri atti di guerriglia urbana non debbono avere alcuna cittadinanza nella nostra società e coloro che lì compiono debbono essere severamente puniti.

A tutte le Forze dell'ordine la nostra solidarietà, particolarmente in un momento così difficile. Onorevoli colleghi, l'ho già fatto indirizzando a nome mio e dell'Assemblea del Senato un telegramma alla famiglia, ma è con profonda commozione che voglio ricordare la scomparsa della senatrice Giglia Tedesco Tatò, figura di primo piano di quest'Aula parlamentare, di cui è stata Vice presidente nella IX legislatura. A nome del Senato della Repubblica e mio personale, desidero quest'oggi rinnovare ai suoi familiari il sincero e profondo cordoglio. Giglia Tedesco Tatò è stata una figura di spicco della vita democratica del nostro Paese fin dall'immediato dopoguerra ed ha posto sempre al centro della sua riflessione ed azione politica l'affermazione dei diritti delle persone, il miglioramento della condizione femminile, la tutela delle minoranze, nella prospettiva del progresso morale e civile della Repubblica. Fu protagonista di battaglie non facili e si schierò con determinazione e generosità, senza mai nascondere i suoi ideali, frutto di una concezione alta e forte della politica. La missione della sua vita è stata proprio questa, la lotta per l'emancipazione e l'uguaglianza delle donne e degli uomini contro lo sfruttamento ed il degrado, nella prospettiva solidale di un rinnovamento della convivenza civile, dove ciascuno potesse sentirsi a pieno titolo cittadino libero e protagonista del proprio destino.

e non solo per ricordarla all'Aula del Senato, ma anche, lasciatemelo dire, per ricordarla a ciascuno di noi, a chi l'ha conosciuta ed a chi ha conosciuto la sua attività

e che pensava che la politica servisse a cambiare il mondo ed a cambiarlo in meglio. Attraverso quell'esperienza si era avvicinata al PCI. Come potremmo però parlare di Giglia se non parlassimo anche del suo impegno a favore delle donne, della sua straordinaria curiosità intellettuale e politica nei confronti delle donne? Lei era una donna cattolica iscritta al PCI, che seppe tessere con il femminismo italiano che seppe tessere con il femminismo italiano e con le organizzazioni delle donne, cattoliche e laiche, un vincolo molto stretto ed appassionato. Stupiva di Giglia la capacità, così lontana dall'archetipo della funzionaria di partito,

per essere classe dirigente, per essere capaci di far crescere il Paese. Dicevo della sua capacità di cogliere l'innovazione. Non c'è stato momento o passaggio nella storia del suo partito nel quale Giglia Tedesco non sia stata capace di essere dalla parte dell'innovazione e del cambiamento, mettendosi in gioco e mettendo pienamente in gioco anche la propria cultura politica, che era fondata soprattutto sulla capacità dialogica, sull'ascolto, sulla comprensione delle ragioni altrui, sulla ricerca del bene comune. fu protagonista di tutte le grandi battaglie di emancipazione delle donne e delle grandi conquiste sui diritti civili e sui diritti delle donne, che oggi fanno parte del nostro sistema, consacrate nei nostri codici. la videro protagonista intelligente, competente e colta, perché fu anche donna delle istituzioni. Alcuni di voi ebbero la possibilità, come il presidente Cossiga, di conoscerla nell'esercizio delle sue funzioni, nella sua capacità straordinaria di essere anche Vice presidente del Senato. Era una donna schiva e riservata, ma era anche molto allegra, ironica, di quella intelligenza che riesce a cogliere nei fatti della vita il lato che ti aiuta a considerarli e a valutarli per quello che sono. Recentemente, da ultimo, è stata pubblicata una sua intervista, curata da Anna Maria Riviello. proprio con le parole di Giglia. «Ho imparato tre cose» diceva «dal PCI ho imparato che il noi è più importante dell'io. Da mio marito, Tonino Tatò, ho imparato che bisogna guardare al futuro, alle cose che bisogna fare. Dal movimento delle donne che bisogna sempre partire dalla propria esperienza, che è una risorsa insostituibile». Credo che queste cose imparate da Giglia passino nella sua lezione anche come eredità nostra e credo altresì che non conti molto l'appartenenza se queste sono, ed è così, le parole di una dirigente politica appassionata alle cose del proprio Paese,

spero che lei e l'Aula mi permetterete di ricordare quella che è stata una mia preziosa collaboratrice quando ero Presidente del Senato, e che, prima di essere mia preziosa collaboratrice, aveva militato, se non nello stesso partito, nelle stesse organizzazioni universitarie cattoliche nelle quali io avevo militato. Giglia Tedesco, moglie di un altro mio caro amico, cattolico-comunista anche lui, cresciuta alla grande scuola dei cattolici comunisti e della sinistra cristiana di Franco Rodano, cattolici veri e comunisti veri, non catto-comunisti (perché non si può paragonare il loglio al grano), ha dato una testimonianza di come si possa vivere con libertà e laicità e la propria fede cattolica e il proprio credo di libertà e di progresso. Signor Presidente, mi auguro che i cattolici del Partito Democratico abbiano la stessa dirittura morale che hanno avuto nel Partito Comunista Tatò e Giglia Tedesco. Presidente, sollecito il Governo perché risponda all'interpellanza da me presentata e pubblicata, atto di sindacato ispettivo 2-00254, pubblicata nel bollettino del Senato, resoconti dei lavori della seduta n. 242 del 6 novembre 2007, con la quale chiedo al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e della difesa, di sapere se il Governo della Repubblica si dichiarerà,

il nostro Gruppo si riconosce nelle parole commosse che lei ha pronunciato per ricordare il tragico sacrificio dei nostri militari a Nasiriya nel corso di una guerra ingiusta dalla quale saggiamente l'Italia è uscita. Ci riconosciamo anche nelle parole di condanna per i gravi fatti di ieri, che hanno visto stroncata una giovane vita e messo a ferro e fuoco interi quartieri della città. E poi un ricordo di Giglia Tedesco. Ho conosciuto Giglia Tedesco da vicino, per un lungo tratto abbiamo militato nello stesso partito, anch'io quel partito l'ho rappresentato in Parlamento, erano gli anni Settanta, anni cruciali della seconda metà del secolo scorso. Conservo molti ricordi di quel periodo, il più bello e vivo è legato alla festa a cui in tante partecipammo all'indomani delle elezioni politiche del giugno 1976, dopo che il Parlamento, grazie a quel voto, era diventato un po' più donna. Giglia Tedesco ha dedicato le sue energie, con l'intelligenza e la *verve* che la contraddistinguevano, a tante battaglie di libertà, democrazia e giustizia sociale, facendo sempre valere in ognuna il punto di vista delle donne. Un impegno particolare lo attivò per la conquista di una maggiore presenza femminile in Parlamento, affermando che la più alta istituzione della democrazia non potesse non rispecchiare e non misurarsi con i nuovi fermenti e i nuovi segni dei tempi; la nuova coscienza e il nuovo senso di sé delle donne erano da annoverarsi tra questi. Dopo i ripiegamenti verificatisi nei decenni scorsi, che condizionano pesantemente anche questo primo scorcio del nuovo secolo, la battaglia per il riequilibrio della rappresentanza di genere è una battaglia ancora tutta da combattere. Anche in nome della senatrice Giglia Tedesco. misurate e commosse parole che lei ha prima indirizzato al Senato e, credo, al Paese intero. Vogliamo soltanto aggiungere alcune riflessioni per esprimere un doppio cordoglio per delle vittime innocenti, anche se cadute in circostanze assai diverse, ma un anche sentimento di indignazione. Non possiamo dimenticare e non dimenticheremo mai i caduti di Nasiriya, che esprimono la parte migliore del Paese, la parte del Paese che sente l'attaccamento al dovere, che sente il senso dell'onore, che sente il compito di portare avanti la propria missione al di là anche della propria incolumità. Vorrei solo ricordare che non caddero per un atto di guerra, ma per un vile e vigliacco atto di terrorismo. Esprimiamo cordoglio anche per quel giovane che, probabilmente estraneo a quello che è accaduto, per un destino veramente incredibile, per le circostanze in cui tutto ciò è avvenuto, ha perso la vita. Vi sono ancora molti lati oscuri in questa vicenda, auspico vicenda, auspico che la magistratura possa fare luce pienamente su quanto è accaduto e anche che, se ci sono delle responsabilità, qualsiasi esse siano, siano punite, come credo il sentimento di civiltà giuridica che il Paese esprime richieda; ma non posso neanche esimermi dall'esprimere l'indignazione per quella parte minoritaria ma tollerata del Paese che si sente in diritto di mettere a ferro e fuoco le nostre città, questa volta per questioni pseudo-sportive, altre volte per questioni di natura politica. Per quanto ci riguarda, per quanto riguarda il mio Gruppo, per quanto riguarda gli elettori e i cittadini che noi rappresentiamo, siamo stufi di questa gente. Auspichiamo un Paese in cui tutto ciò non debba più accadere e nel quale, qualora accada, i responsabili vengano puniti

se qualcuno compie degli atti di barbarie, degli atti che alcune volte sfiorano il terrorismo, degli atti di devastazione, deve essere tollerato.

e riusciremo a reprimere queste manifestazioni, questo sarà il modo migliore per onorare, non a parole ma con i fatti, i caduti di Nasiriya.

una riflessione pur breve. Voglio ricordare Giglia Tedesco, la cui morte ci ha colti tutti di sorpresa - se ne è andata in silenzio e senza volere funerali ufficiali - non solo per quello che è stata, una figura storica, una maestra, un simbolo della storia dell'emancipazione e della liberazione delle donne, della storia del Partito Comunista prima e del PDS dopo. una donna che irradiava forza, simpatia, libertà, amicizia e che parlava a 360 gradi alle donne di tante generazioni e di tante culture. Voglio associarmi brevemente al ricordo di Giglia per dire - la senatrice che mi ha preceduto l'ha giustamente chiamata maestra di innovazione - ciò che era ancora e non ciò che era stata. Dal 2001 Giglia Tedesco, non più giovanissima, si mise convintamente, insieme ai giovani, ai meno giovani, ai circoli dell'Ulivo, a gente nuova, a compagni del suo partito, del suo partito, a capo di un movimento di opinione, di un'organizzazione, dentro e fuori le forze politiche costituite, per l'Ulivo, per i Comitati dell'Ulivo, per il Partito Democratico, testimoniando - lei, lei, che era stata dirigente di un grande storico partito - una curiosità, una capacità di innovazione, di autosuperamento, di stimolo, che certe volte sfidava le più fresche forze di noi un po' più giovani. Giglia Tedesco - lei forse si ricorderà, signor Presidente - affettuosamente insistette negli ultimi mesi, anche con il suo Ufficio di Presidenza, aiutando un collettivo di senatrici, che qui si era fatto promotore, affinché il 2007 fosse celebrato anche in Senato, con la partecipazione di tutte le ex senatrici, come anno delle pari opportunità e dei diritti per tutte e per tutti, rivendicando ancora a sé e al suo lavoro una capacità di proposta e di presenza che non si era mai attenuata negli anni. Giglia Tedesco, specialmente con il suo lavoro negli anni Ottanta e con una riflessione continua sui problemi delle odierne forme di violenza contro le donne e delle nuove tematiche dei diritti, ha testimoniato come la straordinaria stagione degli anni Settanta e Ottanta (che ha aperto al Paese opportunità di diritti, di crescita e di libertà) sempre fosse stata coniugata, nella sua esperienza e nella sua lezione, e potesse esserlo ancora, ai diritti di libertà e di responsabilità collettiva

tutto ciò che in termini di diritti e di opportunità si approfondiva teoricamente: approfondimento teorico, ricerca, ma, poi, inesausta capacità di far legge, di far costume, di operare. Questa è la lezione che, secondo me, modestamente, una generazione di donne, come quella a cui Giglia appartenne, consegna alle generazioni più giovani e che certo ci sfida, perché, accanto a tanta capacità di riflessione, ancora sul tema dei diritti e delle pari opportunità le nostre capacità di far legge e di fare proposta non reggono a livello operativo alla generazione che ci precedette. Signor Presidente, è arduo iniziare una seduta dei nostri lavori con tre commemorazioni su lutti così diversi, ma che tutti ci colpiscono personalmente e politicamente. Per ricordare i morti di Nasiriya vorrei rammentare a me e a tutti voi, senatori e senatrici, che il modo migliore è continuare tenacemente, con ostinazione, a perseguire la politica della pace, a far sì che il nostro Paese non sia coinvolto nelle guerre. Stamattina, uscendo di casa per recarmi al Senato, sono passata in via Attilio Friggeri, dove lavorava Gabriele Sandri. La sua famiglia abita nella strada parallela alla mia e il caffè dove mi reco spesso con mio marito è quello da lui frequentato, probabilmente l'ho incontrato più di una volta. Non posso nascondere il turbamento nel parlare di una vita stroncata a 28 anni in un modo così assurdo, così incomprensibile per me.

Noi - intendendo le istituzioni dello Stato - autorizziamo alcune persone a portare armi e ad usarle in determinate e precise circostanze. Senza nulla togliere alla responsabilità personale di chi stronca una vita - e non entro nel merito del giudizio, non esprimo nessun giudizio - abbiamo una responsabilità politica e istituzionale nel far sì che siano accertate verità e responsabilità,

in quella giornata, dopo quell'episodio, le partite: questa doveva essere una decisione politica. Manifesto il mio dolore personale oltre che politico per la scomparsa di Giglia Tedesco, con la quale ho avuto il privilegio di lavorare, pressoché quotidianamente per cinque anni, in quella esperienza difficile ma appassionante che è stata la Carta delle donne, promossa da Livia Turco e nella quale io e Giglia abbiamo lavorato insieme nella rivista "Reti". Nell'ultimo numero della rivista Giglia, che era contraria alla sua chiusura (decisione che avevamo preso insieme collettivamente),

allo studio e alla ricerca - che Giglia perseguiva - delle cause per cui oggi la libertà e la soggettività delle donne è ancora colpita. In conclusione, voglio ricordare che Giglia era una comunista dell'UDI

tra emancipazione e libertà, tra parità e differenza e, infine, tra appartenenza politica e appartenenza al movimento delle donne. «Non fuggiremo davanti a loro, anzi, li fronteggeremo con tutto il coraggio, l'energia e la determinazione di cui siamo capaci. Ma non li odieremo, anzi, non ci stancheremo di sforzarci di far loro capire che tutto l'impegno dell'Italia, compreso il suo coinvolgimento militare, è orientato a salvaguardare e a promuovere una convivenza umana in cui ci siano spazio e dignità per ogni popolo, cultura e religione». Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo è uno dei passi più significativi dell'omelia che il cardinal Ruini, il 18 novembre 2003, pronunciò in occasione dei funerali di Stato, nella Basilica di San Paolo a Roma, per i tredici carabinieri, i quattro militari e i due civili italiani caduti in Iraq. Nelle ore precedenti quei funerali, migliaia e migliaia di italiani erano saliti all'Altare della Patria, restando in fila per ore, per rendere omaggio alle salme dei caduti e a sottolineare la concreta vicinanza dell'intera Nazione, ma anche la partecipazione della ragione ultima di quel sacrificio. È stata l'occasione nella quale tutti hanno sentito l'unità nazionale come un dato non virtuale, ma concreto e reale. Non so, Presidente, se su questi temi come sul tema della sicurezza di ognuno di noi - oggi sia ingenuo sperare che si recuperi quel comune sentire. Può darsi che sia ingenuo, ma è certamente doveroso; tanto più doveroso, quanto più le nostre forze di polizia sembrano essere diventate dei bersagli. Quel sentire comune di quattro anni fa esige responsabilità, equilibrio e capacità di distinguere. Attendiamo dal Governo, nei tempi più rapidi, una ricostruzione trasparente e completa dei fatti che hanno portato all'omicidio del giovane Sandri. Attendiamo che le responsabilità siano accertate e sanzionate, ma non possiamo accettare quanto accaduto e il fatto che diventi licenza di aggressione nei confronti dei poliziotti da parte dei criminali e dei teppisti. Questa mattina, signor Presidente, ho avuto occasione, per qualche istante, di entrare nella caserma delle volanti di via Guido Reni: ho visto i buchi nei cristalli spessi centimetri provocati dai picconi; ho visto gli occhi smarriti dei rappresentanti della nostra Polizia di Stato, smarriti eppure decisi a continuare nell'adempimento del loro dovere. Un tale smarrimento e simili devastazioni, signor Presidente, non sono degne di un Paese civile. Alla fine, non è un caso che oggi ci troviamo a commemorare la memoria di Nasiriya, a riflettere su quanto è accaduto ieri e a rendere omaggio alla memoria di un illustre parlamentare. Alleanza Nazionale si associa al ricordo della senatrice Giglia Tedesco Tatò. Ogni morte merita silenzio e riflessione: la morte di chi ha servito le istituzioni nelle Aule del Parlamento (come ha fatto la senatrice Tedesco Tatò), la morte di chi l'ha incontrata in una missione di pace la morte banale e tragica incrociata ai bordi di un'autostrada. Nessuna morte va strumentalizzata o messa all'incasso di un partito o di uno schieramento politico. Quattro anni fa, il vicario di Roma parlò dell'Italia in modo toccante, parlò della nostra amata patria, con ciò stesso richiamando il dovere di amarla, intendendo per amore non un sentimento vago, frutto di sensibilità soggettive e mutevoli, ma qualcosa che rimanda a quella giustizia di cui la pietà è una parte. Cicerone ci insegnava che la pietà è l'esatto adempimento dei nostri doveri e che essa raggiunge il massimo verso la patria. Nella fase storica successiva all'11 settembre, e alla sua versione italiana, che è stata Nasiriya, il dovere di amare la nostra patria ha riscoperto radici antiche e frutti nuovi. Anche per questo siamo grati a quei caduti.

Nonostante la circostanza casuale che ha portato a queste commemorazioni, mi sono sforzato di cogliere un elemento comune, un elemento al quale il Gruppo dell'UDC tiene particolarmente. Noi ricordiamo tutte e tre le circostanze importanti alle quali ha fatto riferimento il presidente Marini, esattamente nei termini in cui lui le ha ricordate. Non vorremmo però che, per ragioni di strumentalità di parte, si ricordasse l'una, l'altra o l'altra ancora, a seconda delle proprie posizioni politiche. Noi lavoriamo e continueremo a lavorare perché su queste straordinarie vicende si giunga ad una intesa comune di valutazione dei fatti. Così non è stato per i morti di Nasiriya, ancora stamani. Noi vorremmo che sui morti di Nasiriya si sapesse distinguere tra ciò che ci ha diviso sulla guerra in Iraq, ciò che ci ha distinti sulla nostra presenza in Iraq e ciò che invece ci deve vedere uniti nel ricordo dei nostri martiri. Questa è una grande questione di dignità costituzionale nei confronti della quale stentiamo ad essere - come invece dovremmo - completamente insieme. a Giglia Tedesco, anch'io ricordo con grande piacere di averla conosciuta, in particolare, negli anni della presidenza Cossiga; diaverla conosciuta da cattolica fortemente impegnata in quelle che erano occasioni strettamente di fede che il presidente Cossiga intendeva svolgere al Quirinale, le messe di Natale e non solo, alle quali partecipava da cattolica. Ovviamente da comunista continuava nelle sue battaglie che erano diverse da quelle di essere cattolica. Lei non ha mai ritenuto che si fosse comunisti in quanto cattolici né che si fosse comunisti nonostante si fosse cattolici. Ha saputo essere l'una e l'altra cosa integralmente bene, come è opportuno si sappia fare per evitare che su questo terreno si continuino si continuino ad alimentare pregiudizi a favore dell'una o dell'altra delle questioni. Per quanto riguarda la drammatica morte di ieri del giovane tifoso della Lazio, anche in della Lazio, anche in questo caso non c'è alcuna possibilità se non quella di distinguere la vicenda strettamente calcistica, che richiede accertamenti di responsabilità civili e penali nei confronti di una persona che sembra non avere in alcun modo dato luogo a risse tra tifosi di squadre diverse, da ciò che è avvenuto dopo sua uccisione. Sono cose molto complicate, sulle quali non vorrei che si scadesse, né in una tentazione anti Polizia di Stato, in parte modello G8, né in una tentazione a favore della Polizia di Stato alla quale sarebbe consentito tutto.

possa ancora una volta essere testimoniato come un fatto privato di fede. No, è un fatto di grande rilievo pubblico per il ricordo che il Senato fa di questi tre straordinari avvenimenti molto diversi tra loro; è soprattutto un impegno che il Gruppo dell'UDC vorrebbe ci accomunasse tutti - cosa che ancora non è

Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo della Sinistra Democratica si riconosce pienamente nelle parole con le quali il Presidente del Senato ha ricordato le vittime di Nasiriya. Quali che possano essere i giudizi, le valutazioni sulle scelte di politica internazionale e sulle missioni all'estero, nel momento in cui i nostri militari sono all'estero, su mandato del Governo, qualunque esso sia, e del Parlamento, accanto a loro devono essere - e sono - la Nazione e tutto il Parlamento perché essi svolgono con grande dignità, professionalità, senso del dovere e coraggio i compiti che gli sono stati affidati dall'Italia intera.

Intanto, siamo vicini a lui e alla sua famiglia per il dramma di una giovane vittima che si è spenta. Voglio anche aggiungere le mie parole di solidarietà per le forze dell'ordine che ieri a Roma sono state aggredite in modo indecoroso da gruppi di facinorosi circolanti liberamente per la città. Infine, ricordo anch'io Giglia Tedesco. Ho avuto la fortuna di condividere per due anni l'esperienza senatoriale con lei. Tante cose Tante cose sono state dette di lei e non voglio aggiungerne altre. È stata una delle grandi dirigenti donne della sinistra italiana, che tanto hanno contribuito nel corso del Novecento ad avvicinare le donne alle istituzioni e a consentire alla sinistra politica italiana di coniugare insieme grandi ideali, grande tensione morale e la capacità di affrontare in modo serio, concreto e rigoroso la sfida delle scelte quotidiane. A Giglia Tedesco e ai suoi familiari, va il ricordo affettuoso e la solidarietà delle senatrici e dei senatori della Sinistra Democratica. Signor Presidente, onorevoli colleghi, condividiamo totalmente le parole da lei poc'anzi pronunciate in memoria dei nostri caduti di Nasiriya. Ci uniamo al ricordo della senatrice Giglia Tedesco con profondo rispetto e ammirazione per la sua lunga e feconda esperienza politica. Quanto ai fatti di ieri, vogliamo dire subito che consideriamo la morte di Gabriele Sandri come una sconfitta per tutti: per tutti: per lo Stato, per le forze dell'ordine, per le istituzioni sportive e per il mondo dello spettacolo calcistico. È perciò necessario che tutti ci fermiamo a riflettere, rifiutando letture partigiane e fuorvianti di questa dolorosa vicenda. C'è, innanzitutto, da dipanare la matassa di fatti ancora confusi e di emozioni ancora troppo accese per riprendere il filo della verità: la verità delle cause scatenanti della violenza calcistica, la verità sui mezzi legislativi e organizzativi necessari per fronteggiare efficacemente Ci riserviamo anche noi di ascoltare il Ministro dell'interno. Tuttavia, avvertiamo fin d'ora la necessità di non sottovalutare, per nessun verso e in alcun modo, i fatti di ieri. Esistono oggi, in Italia, almeno 80.000 tifosi estremi, che hanno fatto della violenza uno strumento di ordinaria tifoseria politica e, sempre più spesso, di lotta politica. alcuni gruppi, nelle curve degli stadi, il cui scopo fondamentale è di dirottare la tifoseria estrema verso esiti violenti. La violenza scatenatasi ieri, specialmente a Roma, era preordinata e condotta con tecniche da guerriglia urbana. Ieri sono accaduti fatti che non hanno precedenti nella storia repubblicana e che debbono inquietarci seriamente. Ci auguriamo che venga fatta piena luce sulla responsabilità degli uomini della Polizia di Stato coinvolti nella tragica vicenda di ieri. Ma contro le parole di odio che si sono alzate e che ancora oggi si alzano nei loro confronti, vogliamo ribadire tutto il nostro sostegno, tutta la nostra solidarietà, ben conoscendo i sacrifici che le donne e gli uomini delle forze dell'ordine compiono ogni giorno al servizio della sicurezza e dell'ordine democratico nel nostro Paese.

Signor Presidente, colleghi senatori, anche il Gruppo della Destra ritiene doveroso porgere omaggio, nel quarto anniversario della strage di Nasiriya, ai 19 caduti - ai 12 carabinieri, ai 5 militari e ai 2 civili - che hanno onorato con il loro sacrificio la patria. Era la mattina del 12 novembre 2003 e ancora tutti noi portiamo scolpito quell'agghiacciante episodio che resterà indelebile nei nostri cuori e nelle nostre menti, a perenne memoria del valore e dell'onore degli italiani fuori Patria. Vogliamo inchinarci alla memoria dei nostri fratelli e al dolore delle loro famiglie. Vogliamo poi esprimere la nostra partecipazione al lutto della famiglia del giovane tragicamente caduto e nel contempo portare la nostra piena solidarietà alle forze di polizia che, per uno sciagurato,

fermamente sostenere che occorre tolleranza zero nei confronti di chi attacca uomini, luoghi e simboli delle istituzioni partendo dal presupposto di un tragico evento. Ci inchiniamo al lutto della famiglia Sandri ma, con altrettanta forza,

per la morte del giovane Gabriele Sandri e per la commemorazione della strage di Nasiriya. Aggiungo alle sue parole, signor Presidente, una breve considerazione per la senatrice Giglia Tedesco, che è stata mia grande amica personale. Voglio ricordare le sue doti personali, il suo straordinario temperamento, la sua quotidiana e continua allegria, la sua grande vivacità intellettuale e soprattutto la grande generosità di sé che la rendeva così eccezionale come donna oltre che come politica. Voglio poi partecipare tutta la vicinanza del Gruppo dell'Ulivo alla famiglia di Gabriele Sandri. La sua è una morte assurda, atroce sulla quale chiediamo venga fatta chiarezza e anzi chiediamo di più: che venga conosciuta la verità. Vorrei poi pronunciare due parole sugli episodi di squadrismo vicini alla guerriglia che ieri hanno infangato Roma e altre città del nostro Paese. che la democrazia è tale se è forte e una democrazia forte non può tollerare episodi di questo genere. Dobbiamo chiedere fermezza nel controllo e nella repressione di questi atti vicini alla sommossa, di questi *raid*, di queste aggressioni alle forze dell'ordine: lo dobbiamo fare perché ce lo chiede il nostro ordinamento e, prima ancora, perché è un'esigenza della nostra democrazia. Ha già detto bene lei, signor Presidente, quanto necessario per ricordare il significato della nostra missione a Nasiriya, menzionando il servizio ed il valore, non solo militare, ma anche civile, del sacrificio di 19 italiani. Mi permetta soltanto di aggiungere il ricordo di tutti loro, non solo come militari e civili, ma anche come persone; mi permetta di ricordare che sono morti i Carabinieri sottotenente Giovanni Cavallaro, il sottotenente Enzo Fregosi, il sottotenente Filippo Merlino, il sottotenente Alfonso Trincone, il maresciallo Massimiliano Bruno, il maresciallo Alfio Ragazzi, il maresciallo Daniele Ghione, il brigadiere Giuseppe Coletta, il brigadiere Ivan Ghitti, il vice brigadiere Domenico Intravaia, l'appuntato Horatio Majorana, l'appuntato Andrea Filippa ed i militari dell'Esercito, capitano Massimo Ficuciello, il maresciallo capo Silvio Olla, il caporal maggiore Emanuele Ferraro, il caporal maggiore Alessandro Carrisi, il caporal maggiore Pietro Petrucci ed i civili Stefano Rolla e Marco Beci. *(Generali applausi).* Ricordo i loro nomi perché voglio commemorarli per il servizio che hanno reso, ma anche come persone e come italiani.

colleghi. Vorrei però differenziarmi sulla questione dei fatti di ieri: personalmente, sento il dovere di esprimere una profonda critica ai gruppi dirigenti della Federcalcio.

intervenire per sottolineare la nostra disinformazione: è un fatto gravissimo che per ben dieci ore

che, invece di calmare gli animi, probabilmente li ha accessi ancora di più. Ecco perché ritengo che qui, in quest'Aula, bisogna ricordare questo ragazzo, innamorato della Lazio e della musica, sempre estraneo a qualsiasi violenza, che quindi non ha nulla in comune con i teppisti che volevano commemorarlo con i loro atti di violenza: questo ragazzo generoso, impegnato politicamente e moderato, aveva studiato, si era laureato e, pur essendo benestante, lavorava per crearsi un futuro in piena autonomia.

finestra"). Comunico all'Assemblea che è prevista la presenza in Aula del Ministro dell'interno nel pomeriggio di mercoledì, nel periodo in cui possiamo prevedere, rispetto ai nostri lavori, la sospensione per la Nota di variazioni che deve essere approvata dal Governo per poi passare all'esame

Si tratta di dipendenti degli enti locali comandati presso gli uffici del giudice di pace da diversi anni, ma è evidente che la norma ha un onere molto significativo. Quindi, con un ordine del giorno che poniamo all'attenzione del Governo si potrà nel futuro affrontare questo problema.

deceduti a causa di azioni criminose. Mi rimetto al Governo su questo emendamento. Ove il Governo dovesse essere di avviso contrario, inviterei comunque i proponenti a presentare un ordine del giorno, anche se, in ogni caso, la copertura non sarebbe adeguata.

per cercare di riformulare la disciplina di questa materia, così come vi sono anche altri provvedimenti in tema di vittime del dovere. Pertanto, l'invito è quello a formulare un ordine del giorno, in modo che si possa

Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 24.0.3,

del Corpo forestale dello Stato. Il relatore forse ricorderà che abbiamo avuto modo di parlarne venerdì. In realtà, si tratta semplicemente di un'armonizzazione degli scatti di carriera che non comporta assolutamente alcun onere

almeno chi conosce le vicende del Corpo forestale dello Stato e la necessaria sua equiparazione alle altre Forze di polizia, non possono che condividere l'emendamento meritevole del collega De Angelis. Mentre ho rilevato un atteggiamento di attenzione da parte del senatore Legnini,

Signor Presidente, questo emendamento si riferisce alla necessità, che è sotto gli occhi di tutti - ne abbiamo parlato all'inizio di questa seduta - di adeguare le forze dell'ordine soprattutto per quanto riguarda i mezzi e ancora di più l'organico. Con questo emendamento si tenta di colmare la grave carenza d'organico che c'è nell'Arma dei carabinieri; credo che l'Assemblea dovrebbe prenderlo in considerazione, soprattutto se vuole dare seguito alle tante parole che si dicono

questo emendamento, che propone un risarcimento, una speciale elargizione di 100.000 euro per le famiglie dei sindaci deceduti a seguito e a causa di azioni criminose perpetrate nell'esercizio delle proprie funzioni. È un emendamento costruito su dei fatti accaduti in tempi relativamente recenti, che però ci deve far pensare che i sindaci ricevono giornalmente

Questo è un segnale dal costo veramente limitato. PRESIDENTE. Senatore Rossi, per cortesia, il senatore Franco Paolo sta parlando con il relatore, che invece parla con lei; credo che se poi, si dovranno dare delle risposte, sarà difficile.

rilevante sulle casse dell'erario, vista la modestia dell'importo - a chi è quotidianamente sul fronte, a contatto diretto con i cittadini e spesso purtroppo, come nel caso di un sindaco veneto che è stato ucciso da un dipendente preso da una tensione personale che ha rivolto nei confronti del primo cittadino, ha provocato addirittura un lutto di queste dimensioni. Un voto favorevole non sarebbe assolutamente contrario allo spirito di riconoscimento dell'importante lavoro dei sindaci, di destra o di sinistra, del nostro Paese. *(Applausi dal Gruppo

per la lentezza con la quale procede su questo fronte, che già l'anno scorso venne presentato il medesimo emendamento a pochi mesi di distanza dalla scomparsa di questo giovane sindaco, che ha perso la vita in una situazione straordinaria, che mai si era verificata nel nostro Paese, cioè per mano di un dipendente del Comune improvvisamente impazzito, che ha ucciso il sindaco nel suo ufficio e si è tolto la vita immediatamente dopo. Una tragedia come purtroppo può capitare a chi svolge una funzione delicata come quella di sindaco nel nostro Paese, ma che mai si era verificata in queste particolarissime condizioni. Vista anche l'esiguità della cifra, non credo che sia così difficile trovare una soluzione, signor Presidente, e spiace vedere questo Governo attardarsi e perdere sempre tempo di fronte alle questioni, piccole o grandi che siano, ma che segnano l'attenzione nei confronti dei cittadini.

varrebbe per qualsiasi sindaco, perché si tratta di un sindaco della provincia di Verona, la stessa Provincia del Sottosegretario; credo che un minimo di attenzione da parte del Governo sia almeno doverosa, a prescindere dalle Province dove questo avviene. Mi pare, invece, che il sottosegretario Sartor affronti in modo burocratico questa questione, dimenticando che spesso, al posto dei suoi aridi numeri, ci sono persone in carne ed ossa, con un'anima, un cuore e un'intelligenza. A noi, purtroppo, per la nostra intelligenza, resta solo l'amarezza di prendere atto del fatto che per due anni questo Governo non è riuscito ad affrontare questo banale problema, per il quale chiediamo un po' di giustizia e di attenzione.

Signor Presidente, mi atterrò naturalmente alle indicazioni della maggioranza nella votazione di questo emendamento, mi permetto anch'io di sottolineare la necessità di trovare una soluzione alla singolarità di questa situazione, in cui amministratori pubblici, che rappresentano le istituzioni, sono

la previsione dell'istituzione di un nuovo capitolo nel bilancio del Ministero dell'interno, destinato al rinnovo e all'ammodernamento degli automezzi e degli aeromobili delle forze della Polizia di Stato.

scaturisce però da una ricerca analitica di quello che si poteva raschiare nel nostro barile. Al secondo comma del nostro emendamento, che è il comma 1-*ter*, prevediamo lo stanziamento di ulteriori 10 milioni di euro per fare in modo che non vi siano limitazioni alle prestazioni di lavoro straordinario per la Polizia di Stato. Si tratta di un intervento che consente di mantenere, se non incrementare, gli attuali *standard*, attesa la difficoltà di accedere ad ulteriori assunzioni.

Credo, a questo punto, che tutta l'Aula - ripeto - voglia ben volentieri destinare alla Polizia di Stato tali risorse, anche alla luce delle considerazioni che alcuni di noi hanno espresso all'inizio di seduta.

È una piccola goccia nel *mare magnum* di una grande necessità che riguarda le forze di polizia e - aggiungo - anche gli operatori e gli uomini in divisa. Mi sembra ad ogni modo scontato che sia un segnale di buona volontà dell'Aula e che questo emendamento vada in un'ottima direzione.

conforme al relatore.

di ottenere più) un incremento di 10, dico 10 milioni di euro per il 2008, per quanto riguarda i nuovi automezzi (e bisogna sapere di che si tratta, parlando anche degli aeromobili), e di 10 milioni di euro per gli straordinari, e si tratta di capire di Il Gruppo dell'UDC, come il collega Ciccanti dirà dopo, ha proposto ben altra cifra (si tratta di 500 milioni di euro) sull'articolo 93 e quando verrà il momento il senatore Ciccanti illustrerà

che indirettamente con gli emendamenti che propongono articoli aggiuntivi trattano di materia riguardante il potenziamento delle Forze di polizia e delle Forze armate (come abbiamo visto all'articolo 22).

finestra") *(UDC)*. Signor Presidente, so bene che può apparire una forzatura chiedere che non si proceda

Chi vive però in quelle Regioni sa bene che, anche per effetto di normative farraginose e burocratiche, la ricostruzione, ad oggi, non è ancora completata e le ferite dei centri storici e delle frazioni maggiormente colpite sono ancora aperte. Quello che con l'emendamento 27.6, insieme ai colleghi Ciccanti, Forte e Baldassarri, intendiamo chiedere è l'equiparazione, soprattutto per i cittadini umbri e marchigiani, dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi con quelli disposti a favore dei soggetti interessati dal sisma del 1990 verificatosi nei territori delle Province di Ragusa, Siracusa e Catania, oltre che dagli eventi alluvionali nella Regione Piemonte: in questi era stato stabilito che la posizione contributiva fosse regolarizzata con il versamento del 10 per cento dell'importo dovuto. Se dovesse passare senza modifiche l'articolo 27 e dovesse essere bocciato l'emendamento 27.6, sarebbe confermato un principio estremamente pericoloso, e cioè che esiste una disparità di trattamento tra i cittadini italiani e che gli stessi non sono uguali di fronte alle calamità naturali.

istituisce uno specifico programma, presso il Ministero delle risorse agricole e forestali, per un uso corretto delle risorse idriche in agricoltura. Se ne era già discusso in un'altra occasione:

faccio rilevare al collega Turigliatto che questo tema è già stato affrontato e, in parte, risolto con l'emendamento, accolto in Commissione, sul piano irriguo,

Nel DPEF era stato affermato che gli obiettivi da portare avanti per il settore agricolo e agroalimentare erano due: quello della stabilizzazione del trattamento fiscale agevolato per l'agricoltura e quello del rafforzamento dei controlli

ditte che non hanno niente a che vedere con la produzione nazionale, ma che possono fregiarsi di simboli, bandiere e nomi storpiati che ad essa fanno ricondurre molti prodotti.

biomasse e da residui agricoli, una incentivazione molto forte, sia per i certificati verdi che per la tariffa con cui viene stabilito il concambio. Questa agevolazione permette oggi di dare un forte impulso alle agroenergie. Poi sono stati compresi 30 milioni per rifinanziare il fondo di solidarietà nazionale, soldi che servono per pagare

Venendo proprio alla finanziaria, i due temi prima citati, quello della stabilizzazione del trattamento fiscale e quello dei controlli, sono stati ampiamente affrontati e risolti con opportune misure.

a livello europeo; la definizione delle attività forestali come passibili dei benefici del protocollo di Kyoto; la norma sull'apicoltura per un piano di settore; la sospensione delle procedure esecutive per le aziende agricole sarde, in grossa difficoltà per il pignoramento delle proprie aziende; una bella norma sulla trasparenza del mercato, che affronta il problema dell'incremento dei prezzi agroalimentari che tanta parte hanno avuto in quest'ultimo periodo nella ripresa dell'inflazione; infine e qui mi collego all'emendamento del senatore Turigliatto - c'è un rifinanziamento importante del fondo per il settore irriguo con 100 milioni a far data dal 2010. Concludo il mio intervento per dire che questo Governo e questa maggioranza continuano ad avere grande attenzione per il settore agricolo e agroalimentare.

L'attenzione che il Governo Prodi in due anni ha riservato al settore agricolo, per quanto riguarda la stabilizzazione fiscale in agricoltura, è la seguente: è stata reintrodotta la tassa di successione in agricoltura come per gli altri cespiti patrimoniali.

dell'articolo 5 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, del quale non si parla assolutamente nel comma uno dell'articolo.

Presidente, faccio rilevare che, sicuramente, stando al testo dell'articolo, i commi 6 e 7 devono essere votati cumulativamente perché ad essi, cumulativamente, fa riferimento la copertura. Non vi è nessuna possibilità di distinguere quanta parte della copertura sia riferita al comma 6 e quanta al comma 7.

affidato ad una proposta di legge una riforma organica sulle questioni relative alla pesca. Ho preso la parola su questo articolo perché

di sospendere la vendita all'asta delle circa 7.000 aziende - sospendere purtroppo temporaneamente

il finanziamento delle opere previste dal Piano irriguo nazionale e, in generale, sulle misure previste nel disegno di legge finanziaria 2008 a favore del comparto primario, per le quali la 9a Commissione del Senato ha voluto fornire i propri contributi. In primo luogo, l'articolo in esame, che prevede una serie di interventi nel settore dell'irrigazione, riveste notevole importanza, perché fornisce una risposta di tipo strutturale alle problematiche del comparto, in materia di risorse idriche, affrontando il problema della scarsità delle stesse e del loro non razionale utilizzo in agricoltura, consentendo così di superare le emergenze provocate dal fenomeno della siccità. Con il disegno di legge finanziaria all'esame, vengono pertanto previsti finanziamenti per 5 milioni di euro, per ciascuno dei prossimi tre anni, per l'attività di progettazione delle opere irrigue e per la prosecuzione dei lavori già avviati, in già avviati, in base al Piano irriguo nazionale predisposto con la legge finanziaria dello scorso anno. È previsto, inoltre, un ulteriore, consistente contributo di 100 milioni di euro, per la durata di 15 anni a decorrere dal 2011, per il completamento e la definitiva realizzazione di numerose opere contenute nel Piano stesso. Sottolineo, pertanto, che tale tipo di intervento consentirà di realizzare, in tempi che auspico rapidi, le opere già previste dal Piano irriguo nazionale e di avviare prossimamente un secondo Piano irriguo che tenga conto delle esigenze di alcune aree del Paese, come le Regioni meridionali e, in particolare, le isole che, durante la stagione estiva, sono particolarmente colpite dal fenomeno della siccità con gravi conseguenze per tutto il comparto e degli indubbi danni economici per gli imprenditori agricoli. Voglio evidenziare, inoltre, che le misure contenute nella manovra di bilancio si muovono nella direzione richiesta dalla stessa Commissione agricoltura, sia nel corso dell'esame dello scorso Documento di programmazione economico-fìnanziaria, sia nelle osservazioni contenute nel parere reso alla Commissione bilancio sul disegno di legge finanziaria per il 2008. sottolineo, comunque, l'opportunità di continuare a prevedere, oltre a una serie di interventi strutturali, anche delle efficaci misure che consentano una corretta gestione delle risorse idriche, attraverso, ad esempio, la realizzazione di impianti che, utilizzando le moderne tecnologie, consentano un maggior risparmio idrico e una razionalizzazione delle risorse stesse. Ritengo, infine, che la gestione delle risorse idriche, come è emerso in numerose occasioni nel corso dei lavori della Commissione agricoltura

**Il Senato approva.** Passiamo all'articolo 27, Signor Presidente, la proposta di emendamento si inserisce nell'articolo del disegno di legge Finanziaria che incentiva la produzione di energia da fonti rinnovabili, in un'ottica che contempera la tutela ambientale con l'esigenza di superare le note carenze del sistema energetico nazionale. L'emendamento intende quindi eliminare il divieto imposto dalla legge n. 179 del 2002 all'estrazione di idrocarburi in Alto Adriatico in quanto, dalle ricerche che erano già state svolte prima di tale legge, risulta che in tale zona possono trovarsi riserve di idrocarburi il cui sfruttamento, nel rispetto della tutela ambientale - sottolineo - fornirebbe un ulteriore valido ausilio al sistema energetico nazionale. La modifica proposta darebbe in sostanza la possibilità di effettuare l'attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi nella zona dell'Alto Adriatico dopo aver accertato che esse sono compatibili con l'ambiente e, in particolare non sono responsabili del fenomeno della subsidenza ovvero dell'abbassamento della superficie terrestre. In conclusione, mi sembra quindi che in tal modo si contemperi la necessità della salvaguardia ambientale con quella altrettanto importante di sfruttare riserve energetiche fondamentali per il Paese. Faccio presente che non ha evidentemente bisogno di copertura finanziaria; anzi; porterebbe introiti maggiori allo Stato. In ogni caso, chiedo comunque che la votazione sia effettuata con il sistema elettronico.

L'articolo 30 è l'unica norma in tema di missione energia contenuta nel disegno di legge originario; tutto il resto di questo Capo IX è stato aggiunto in sede di Commissione.

dal Governo in occasione della discussione e del voto finale della legge comunitaria. In sostanza,

a fonti diverse dal petrolio ma talvolta di origine petrolifera; sussidi che non assolvono a funzioni

cascami del petrolio ed altre fonti energetiche. Il Il tema è stato anche oggetto di discussioni in sede comunitaria e di contestazioni al nostro Paese. La legge finanziaria dell'anno scorso introdusse una disciplina, in parte transitoria, in parte definitiva; in sostanza, pose termine a quello che da molti era considerato un abuso o addirittura uno scandalo. Ricordo che non era solo

sussidi agli assimilati sembrava si fosse alterato anche il campionato di calcio, consentendo a certe squadre di comprare dei giocatori. Dopo l'approvazione della legge finanziaria nulla è stato fatto dal Governo in attuazione di tale norma. Era stato presentato un articolo correttivo in sede di legge comunitaria, che è stato stralciato

il venir meno del procedimento comunitario e il preciso impegno del Governo, nella persona del ministro Bonino, a ripresentare l'articolo in sede di legge finanziaria.

questioni. L'articolo 30, di per sé, porta finalmente a compimento la riforma del CIP 6 e l'eliminazione della stortura, tutta italiana, che faceva sì che dal 1992 ad oggi le risorse energie rinnovabili fossero attribuite ad impianti che producevano energia certamente non da fonti rinnovabili. Attraverso l'*escamotage* delle fonti assimilate, dal 1992

oggi mettiamo fine, dopo una discussione lunga e articolata, durata quasi un anno, a questa stortura. Contemporaneamente, introduciamo un'altra grande parte della riforma, riguardante gli incentivi per le energie rinnovabili. dopo l'inserimento nel cosiddetto decreto fiscale della riforma degli incentivi sulle biomasse agricole, completa il sistema

consente, quindi, da una parte, di uscire dallo scandalo del CIP 6 e, dall'altra, di recuperare quei fondi destinati alle fonti assimilate per compiere questa operazione di riordino del sistema degli degli incentivi alle energie rinnovabili. Ciò attraverso due meccanismi. Si prevede un meccanismo di certificati verdi per gli impianti al di sopra di un megawatt e un sistema di ritiro a tariffa omnicomprensiva, ossia il cosiddetto conto energia, per gli impianti al di sotto di un megawatt. Soprattutto, finalmente tra le diverse fonti previste dalla direttiva europea sugli incentivi delle fonti rinnovabili, ma in relazione alla sostenibilità ambientale. Non si finanziano quindi le fonti tutte allo stesso modo, ma si fanno delle scelte precise, per cui, da una parte, si incentiva

Paese e la sola possibilità che abbiamo per guardare al futuro con serenità per quanto riguarda l'energia. Ciò al contrario di alcuni dibattiti un po' stantii che continuano a far discutere il nostro Paese su questioni come il nucleare, che guardano al passato e non certamente al futuro e all'innovazione per quanto riguarda le energie rinnovabili. *(Applausi Signor Presidente, onorevoli colleghi, sono consapevole del fatto che il mio Gruppo ha soltanto pochi minuti a disposizione per intervenire. Da sempre

sia stato un modo improprio di considerare le fonti rinnovabili. Non vediamo alcun contrasto tra il riproporre, come noi facciamo, il tema del nucleare, che è una fonte rinnovabile, e le altre fonti rinnovabili. A differenza dei Verdi noi siamo per lo sviluppo e non per il blocco del Paese. *(Applausi

Con questo emendamento autorizziamo anche quei progettati non ancora approvati. Via via le parole hanno un loro senso: eravamo contrari prima e rimaniamo contrari ancora oggi; le poche risorse presenti vanno concentrate sulle fonti rinnovabili.

Signor Presidente, colleghi, contrariamente a quanto dichiarato da alcuni colleghi che vedono nelle energie alternative la possibilità di risolvere il problema energetico del Paese, noi, ahimè, siamo di tutt'altra opinione, di tutt'altro parere. durante il mio primo mandato parlamentare, nel 1994, proprio in questo Senato, c'era un consenso trasversale

Ora mi sembra che si cominci a parlarne abbastanza liberamente, che si cominci ad affrontare il problema, che è un problema reale del Paese.

Contrariamente a quello che ha detto la senatrice poco fa, tutto il mondo sta rivedendo la sua politica nucleare; tutto il mondo è conscio che se non si va verso il nucleare non si risolvono i problemi energetici del Paese. So di dire cose scontate e conosciute, ma voi sapete benissimo da chi compriamo l'energia nucleare: la compriamo dalla Francia, che ha

le disposizioni che sono state date attraverso quel famoso *referendum* che ha abolito il nucleare in Italia sull'onda della tragedia

venire. Ritengo che affrontare lo sviluppo del Paese con le nostre industrie che pagano l'energia elettrica il 30 per cento in più degli altri Paesi sia da incoscienti.

ricordare che proprio oggi è qui a Roma il Segretario del Dipartimento dell'energia degli Stati Uniti per firmare con il ministro Bersani un protocollo di intesa per lo sviluppo della ricerca nel campo nucleare, quella sovvenzionata da questo fondo, per la cosiddetta *Generation IV*, che è la prospettiva di generazione di nuovi impianti nucleari. L'energia nucleare è un bene enorme per l'umanità ed ha un potenziale di sviluppo gigantesco, come sa chiunque la conosca.

è davvero tale da non poter essere rifiutata da qualunque persona di buon senso. Qui si prevede di sviluppare delle ricerche

ai fini della risoluzione dei problemi del caro prezzo delle fonti di energia e quindi del rallentamento o comunque dell'impedimento dello sviluppo delle attività produttive, sia come parlare di qualcosa che sta fra gli obiettivi utopici e la fantatecnica. Cosa è, infatti, parlare di ricerca per l'energia dell'atomo di cosiddetta quarta generazione (ed io do atto al Governo di essere su questa su questa china, su questo indirizzo); altra cosa è parlare, *tout court*, di produzione energetica per via dell'atomo, come fa la Francia o altri Paesi produttori.

tuttavia sottolineare una posizione difforme da quella espressa dal mio collega Stefani, perché perché (innanzi tutto da un punto di vista etico-politico) non credo che sia aderente ad un movimento localista e con radicamento popolare, né ritengo sia di grande interesse parlare di energia nucleare. Non credo che un movimento popolare che deve essere attento anche alle indicazioni popolari

Credo che fare riferimento alle situazioni di produzione di energia attraverso l'atomo attualmente (è il caso della Francia, come diceva il collega Stefani) significa non tener conto che proprio quella produzione di energia è avvenuta a condizioni tecnico-amministrative tali da non poter oggi consentire la privatizzazione

a stare attenti: una cosa è sollecitare le forze parlamentari e i Governi verso la ricerca più approfondita, con mezzi cospicui nella direzione della produzione dell'energia, diversa però da quella che finora e tuttora si produce; una cosa è dare per scontato

ci porterà sulla soglia di una terribile emergenza, che purtroppo è già annunciata. Il problema - lo dico anche in senso autocritico - non si risolve con le mozioni di sfiducia *ad personam*, che io personalmente e molti altri in Parlamento non sottoscriveremo mai.

contenzioso infinito, che arricchirà soltanto gli avvocati, e che la norma è retroattiva al 2007. Pertanto stiamo per approvare un provvedimento che, al di là della sua valenza economica, avrà un pesante influsso sul sul contenzioso. Ripeto, è una norma scritta su dettatura dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Credo che la politica dovrebbe poter dire qualcosa in modo più autonomo.

ai produttori di energia elettrica mediante fonti rinnovabili. Non scendo nel dettaglio, ma stiamo parlando, al 2012, di 4-5 miliardi di euro, un costo aggiuntivo al nostro kilowattora, che è già il più caro d'Europa, dell'ordine del 15-20 per cento. Ma come possiamo, avendo a cuore la competitività del nostro Paese, gravare così tanto sul kilowattora,

L'emendamento 30-*ter*.100 cerca di attenuare, nei limiti del possibile, questa eccessiva incentivazione e questo dirigismo. che la produzione di energia elettrica verrà incrementata dello 0,75 per cento per anno dal 2007 al 2012, che è

ogni tre anni è minima ma, almeno, testimonia una incentivazione che si riduce nel tempo. Non c'è alcun motivo di mantenerla così elevata.

Mentre l'Unione Europea ha aumentato la produzione da fonti rinnovabili dal 1997 al 2005 di 111 terawattora (e sono miliardi di kilowattora), la produzione italiana è rimasta ferma intorno ai 51 terawattora. significa che il nostro sistema d'incentivazione è troppo debole e il nostro sistema autorizzativo troppo complesso. Il Consiglio europeo ha deliberato il 6 marzo, in forma vincolante, l'obiettivo del 20 per cento di energia da fonti rinnovabili nell'Unione Europea Invece, il senatore Possa propone che, per legge, l'incentivo alle fonti rinnovabili diminuisca del 5 per cento ogni tre anni. Nessun Paese europeo applica una norma del genere. Mentre le fonti fossili crescono,

tenendo conto del risparmio di 1,3 miliardi di euro al 2012 per l'eliminazione del CIP 6 in quota alle assimilate non più rinnovabili,

A regime significa 30 milioni di tonnellate di emissioni di CO2in meno: pagheremo cara la CO2 in più rispetto agli obiettivi di Kyoto, per non parlare poi del risparmio in milioni di tonnellate equivalenti di petrolio. Si tratta anche di una buona operazione economica. L'Europa è *leader* mondiale di fonti rinnovabili. Dei 40 miliardi di dollari annui, 15 sono investiti dall'Unione Europea. Il settore delle rinnovabili ha creato in Europa 300.000 posti di lavoro. In Germania, che è *leader* europeo delle rinnovabili, sono 114.000 gli occupati e l'anno scorso gli occupati nel settore delle rinnovabili hanno superato quelli dell'industria automobilistica. Quindi, è un buon investimento economico ed una forma di energia nazionale pulita. Vale la pena di incentivarla riformando il sistema.

fonti rinnovabili in energia elettrica. L'articolo in esame al comma 1, lettera *h)*, prescrive che l'autorizzazione alla realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili non può essere subordinata a misure di compensazione

installazioni di impianti per la trasformazione in energia elettrica di energie rinnovabili, è di ostacolo alla diffusione degli impianti stessi. Ebbene, ho il dovere di riferire all'Aula un'esperienza che va in senso completamente diverso,

la quota più alta nell'uso delle fonti rinnovabili trasformate in energia elettrica. Posso assicurare che ogni autorizzazione è accompagnata da una convenzione, che regola i rapporti fra la società installatrice ed il Comune e prevede

per le altre energie primarie (vedi i pozzi petroliferi), i territori coinvolti ed i Comuni vengano ristorati per l'utilizzo di queste forme di energie alternative.

in questione mi pare particolarmente importante, perché introduce disposizioni che conferiscono risorse consistentissime alle produzioni militari:

mi pare che le risorse siano enormi e che, ancora una volta, di fronte ad un elemento di grande contenutezza, dal punto di vista delle disponibilità verso i settori sociali, vi sia invece grande disponibilità ad aumentare le spese militari.

di Nasiriya e la memoria ci spinge ad onorare i caduti delle missioni di pace, l'Assemblea dovrebbe essere interessata al dibattito, sicuramente molto importante, sollecitato anche dal Presidente della Repubblica di recente con un intervento mirabilissimo sulle spese per la difesa e per la sicurezza dei nostri uomini. Credo che l'Assemblea debba respingere all'unanimità la richiesta del senatore Turigliatto non perché in Aula si discuta di militarismo a tutti i costi, ma perché ormai è tempo che in Italia si costruisca una cultura della difesa e che si dica con chiarezza ai nostri concittadini ed agli italiani tutti che le forze dell'ordine, le forze armate, gli uomini in divisa garantiscono all'estero la sicurezza e la stabilità nei contesti internazionali. Chiediamo a questi uomini, per poche lire al mese ed al costo del sommo sacrificio della vita, la sicurezza nel nostro Paese, fuori di esso e perfino compiti che non sono stati loro istituzionalmente mai indicati come necessari, come quelli della lotta all'abusivismo edilizio in alcuni casi e della realizzazione perfino in casi di emergenza delle discariche, come è accaduto in Campania. Che cosa dobbiamo chiedere di più alle Forze armate, agli uomini in divisa non so! E puntualmente il Governo e l'Assemblea vengono interessati da ragionamenti folli sulla contrazione di un bilancio che non garantisce nemmeno l'ordinaria amministrazione. I Capi di Stato Maggiore ed i comandanti generali si sono già pronunciati all'interno della Commissione difesa. Chiedo all'Assemblea di respingere l'emendamento del senatore Turigliatto all'unanimità per dare un segnale a quei martiri e militari che stanno combattendo all'estero per la nostra sicurezza, dentro e fuori del Paese. È difficile considerare strumento di difesa una cosa che si chiama Eurofighter. Del resto, nel primo intervento in Aula sulla finanziaria, ho appunto detto che abbiamo bisogno di una diversa scrittura del bilancio delle spese militari perché in Commissione difesa arrivano quasi solo le spese di esercizio. Tutti gli investimenti, pesantissimi, avvengono in altre aree, sicché la costruzione, la vendita, la sperimentazione di armi diventa alla fine, come è stato detto da illustri rappresentanti delle industrie che le producono, la colonna del bilancio dello Stato italiano. Non posso accettare che la colonna del bilancio dello Stato siano il piazzamento e la vendita di strumenti di distruzione, anche di massa nel mondo. Abbiamo di recente votato alle Nazioni Unite una mozione contro l'uso dell'uranio. Bisogna mettere un po' di razionalità in questo atteggiamento: tirare di mezzo le emozioni suscitate da Nasiriya è assolutamente strumentale ed incredibile.

che ha firmato l'emendamento, sperando che non se ne dimentichi - e Rossi si ricordino che oggi celebriamo un triste anniversario ed è il giorno più sbagliato per portare all'attenzione dell'Aula questo tipo di argomenti.

politicamente potremmo utilizzare le contraddizioni interne alla maggioranza per arrivare a voti imprevedibili. Ci sta però a cuore la ricerca nel comparto navale, terrestre e militare,

la sinistra non riesce a portare avanti una politica estera oppure no? Qualcuno ha parlato di uranio. Gentile collega, vorrei ricordarle che c'è stato un unico caso in tutta la storia della Repubblica italiana in cui è stata dichiarata una guerra senza che il Parlamento ne fosse AN e UDC).* Oggi ci sono 1.200 soldati, o ex soldati - e qualcuno anche ex essere umano, perché è deceduto - colpiti da malattie legate all'utilizzo di armi all'uranio,

Attenzione, perché allora ci fu un inganno clamoroso in cui siamo caduti tutti; bisogna riscrivere bene quella parte di storia, soprattutto per il futuro. Ma allora, come la mettete, cari colleghi della sinistra? Dove sono le vostre bandiere della pace? Qualcuno oggi, coerentemente, continuerà a sventolarle, ma gli altri?

ad un dilemma che non credo sia così secondario. C'è un problema. Credo che oggi, nell'anniversario dei caduti di Nasiriya, francamente non si possa votare contro le nostre Forze armate. Va sottolineato un dato: ancora una volta quando si tratta di Forze armate e di politica estera questo Governo non ha la maggioranza. Vorrei che se ne ricordasse anche il presidente Napolitano.

dai nostri militari all'estero. Non capisco come si possa non comprendere questo o far finta di non capirlo. Non possiamo nemmeno sacrificare alla ragion politica interna

ideale, politica ed etica, che non vuole più mandare dei soldati italiani in giro per il mondo a farsi uccidere e qualche volta ad uccidere altri. Proprio perché ho molto

e le riduce drasticamente; non le abolisce completamente, ma le riduce drasticamente. Credo che sia esattamente una concezione di pace quella che ispira

che hanno testimoniato fiducia alle nostre Forze armate impegnate in missioni di pace. Quest'Aula ha votato in senso *bipartisan* più volte. Mi piacerebbe sapere chi, in quest'Aula, ritiene che oggi bisogna tagliare i finanziamenti alle Forze armate che garantiscono la politica estera del Paese nel mondo.

in un intervento nel quale esprime un parere politico, attribuire ad altri colleghi espressioni che non sono state

non va visto soltanto, come giustamente è stato espresso, in termini di considerazione o meno delle Forze armate italiane, che a mio parere sono fuori discussione, ma va visto in chiave politica: è un emendamento che francamente non ha nessun senso. Scusate, ma il nostro impegno nelle operazioni di pace è un impegno sotto l'egida delle Nazioni Unite. Voi cosa volete? Vivere fuori dal mondo? Volete che Volete che l'Italia non partecipi ad uno sforzo per portare pace, stabilità, serenità a popolazioni che ne hanno bisogno e identificate questo discorso, ipocritamente e falsamente, come avete sempre fatto, con le balle della guerra che porta anche ad uccidere altri ed altre facezie del genere. Il vostro errore è di non capire che quando si partecipa di una responsabilità di Governo bisogna gestirla responsabilmente e non si possono continuare ad avere

quello che abbiamo fatto per i precedenti emendamenti: non parteciperemo al voto, perché non intendiamo, con il nostro voto, andare in aiuto a questa sinistra che non riesce mai ad uscire dalle contraddizioni ogni volta che si parla di politica estera.

solo per dichiarare l'orgoglio per l'opera dei soldati italiani che difendono la pace nel mondo. Vorrei dire al proponente di questo emendamento che io sono stato in Kosovo, dove i monaci serbi possono vivere perché ci sono i soldati italiani e sono stato commosso dalle attestazioni di gratitudine che sono venute non soltanto dai monaci, ma da tutta la popolazione serba del nord del Kosovo, la Metohija, che sanno di dovere la possibilità di vivere, e di vivere nelle loro case, alla presenza italiana. Vorrei anche ricordare che la Duma la settimana scorsa ha sospeso il Trattato di moratoria sugli armamenti convenzionali in Europa.

certo non mutamenti nel senso di diminuire l'efficienza del nostro strumento militare, che è stato ridotto esattamente quando, dopo il Trattato di moratoria, si arrivò ad una decisione di disarmo comune e bilanciato in Europa.

Voglio però dire qualcosa anche sul modo distorto con cui è stata presentata a quest'Aula la nostra posizione, intanto con un collegamento strumentale e inaccettabile con la tragedia di Nasiriya. Come ho detto poco fa, quando una missione è votata e i militari sono all'estero, essi sono difesi da tutto il Parlamento, ma si ha comunque il sacrosanto diritto di essere contrari alle missioni militari e questo non toglie nulla alla difesa delle nostre Forze armate impegnate all'estero.

Quindi, meno propaganda e più sostanza, per favore!

nel nostro Paese la natalità diminuisce e il numero delle donne lavoratrici autonome aumenta. Alle lavoratrici autonome ad oggi non viene riconosciuto il diritto di vivere serenamente il periodo della gravidanza, dovendo sospendere e rallentare il proprio lavoro ed essendo per di più costrette ad adeguare il proprio reddito ai parametri stabiliti dagli studi di settore anche durante la gravidanza e l'allattamento. Esiste dunque nel nostro Paese una disparità di trattamento tra lavoratrici autonome e lavoratrici dipendenti, che non possiamo più far finta di non vedere. Se volessimo in qualche maniera parafrasare una frase che va di moda in questo periodo, potremmo dire serenamente, ma altrettanto chiaramente, sull'onda di Crozza-Veltroni, che noi siamo per il lavoro, ma siamo anche per la tutela della maternità. Per questo, di fronte al rischio che molte donne, nell'impossibilità di adeguarsi agli studi di settore, lascino il mercato del lavoro ed altre decidano di rinviare sempre di più la gravidanza, invitiamo il Governo,

vale a dire quello della gravidanza sommato al primo anno di vita del bambino.

quasi di contenuto normativo e questa è la ragione per cui invito il Governo ad accoglierlo come raccomandazione.

al problema delle donne lavoratrici autonome a mezzo dell'esclusione dai parametri degli studi di settore andrebbe attentamente valutata: non è detto che sia una soluzione adeguata. Tanto più che l'attuale ordinamento prevede comunque per il contribuente la possibilità di presentare le proprie controdeduzioni e giustificazioni, nel caso in cui non ci si adegui per una ragione fondata agli studi di settore. Pur tuttavia, cogliendo una sensibilità su questo tema, a questo punto, essendo stata manifestata l'insistenza sul voto, mi rimetto all'Assemblea: ciascuno decida come ritiene più opportuno.

ma in un Paese nel quale quello legato al rapporto tra la possibilità di avere figli, le gravidanze e il lavoro femminile è un punto ancora non compiutamente definito, lo considerano comunque un contribuito alla discussione. Questa è la ragione per la quale voteremo a favore.

a cui chiedo di apporre anche la mia firma. Penso che affronti un problema molto importante. Certamente, dal punto di vista del dettaglio e delle modalità sarà poi compito del Governo e di questo Parlamento approfondire questo tema questo tema ed anche risolverlo, perché noi abbiamo a cuore l'autodeterminazione delle donne e quindi il fatto che possano scegliere quando e come diventare madri e poi anche come e quando lavorare.

Presidente, l'ordine del giorno affronta giustamente un tema di grande rilevanza, che riguarda la possibilità per le donne lavoratrici autonome di di accedere alla gravidanza con tutte le garanzie, così come per tutte le altre donne. Tuttavia, nella premessa che, secondo me, non può essere accettato. Sarei disposto a votare questo ordine del giorno se venisse cassato il passaggio che prevede il fatto che molte lavoratrici autonome, dal momento che non si possono adeguare agli studi di settore, escono dal mercato del lavoro. Questa, intanto, mi sembra un'affermazione non dimostrata e comunque sbagliata e contraria alla linea di politica economica del Governo. Chiedo quindi di sopprimere questa parte. Eventualmente, poi, il nostro voto potrebbe essere favorevole. Grazie,

per la ragione che qui si adombra il rischio legato all'impossibilità di adeguarsi agli studi di settore da parte delle donne che vivono la condizione di gravidanza e quindi esiste il rischio reale, proprio per l'incertezza e la particolarità della condizione, di lasciare la propria attività. Non è

assolutamente non condivisibile, in cui si parla di "una evidente disparità tra la condizione delle donne lavoratrici autonome e quella delle lavoratrice dipendenti" sulla maternità. Faccio notare che le lavoratrici dipendenti

La nostra volontà era di votare a favore, ma per un mero disguido tecnico, l'espressione del voto è stata negativa. Vogliamo che ciò rimanga a verbale, perché l'impegno in Commissione, almeno per quanto riguarda il Gruppo UDC, è a favore dell'articolo misure per onestà nei confronti della Commissione bilancio ed anche nei confronti dei cittadini.

attraverso i quali si incentivavano le rotte di trasporto merci, le cosiddette autostrade del mare. Nel primo decreto la Sardegna non veniva nemmeno menzionata, mentre nel secondo venivano inserite nella rete delle autostrade del mare

Si tratta chiaramente di una presa in giro e, in ogni caso, di una palese ingiustizia nei confronti del sistema produttivo sardo e dei trasportatori, della Sardegna e del continente, che non possono usufruire del *bonus* cui usufruiscono gli altri trasportatori nelle altre rotte nazionali. In particolare, per la Sardegna questo è un fatto ancor più grave perché perché le porte di accesso del trasporto merci sono nel Nord dell'isola mentre la maggior densità di insediamenti produttivi e residenziali

Se e vero, come è vero, che le "autostrade del mare" sono state fatte per trasferire una quotadi traffico dalla terra al mare, eliminando i costi di congestione, non si capisce perché le rotte tra la Sardegna

L'emendamento tende pertanto ad includere le rotte sarde nelle "autostrade del mare" e, in questa maniera, ad eliminare un'ulteriore ingiustizia nei confronti della nostra comunità sarda.

si vogliono estendere i finanziamenti previsti per le «autostrade del mare» ai collegamenti con le isole minori. Faccio rilevare che già l'articolo 16 della legge finanziaria contiene una norma

dalle isole minori anche a questa finalità. Per questa ragione, pur affrontando l'emendamento una problematica che merita tutta la nostra attenzione, esprimo parere contrario.

contrario. L'emendamento 34.9 estende i contributi per le imprese che effettuano il trasporto combinato all'asse ferroviario del Corridoio 5 e del Corridoio 1.

intaccato, ove noi dessimo un parere favorevole a finalizzazioni che rischiano di squilibrare l'intero articolato.

all'articolo al nostro esame, alla realizzazione di interventi infrastrutturali per la messa in sicurezza delle strade sulle quali si registrano i più alti tassi di incidentalità. Il problema è molto serio e, peraltro, è già affrontato

34.14, esprimo parere è contrario. Esso intende ridurre risorse destinate alle infrastrutture per destinarle all'edilizia penitenziaria. Come il senatore Caruso e gli altri sanno, questa finanziaria già prevede risorse aggiuntive per l'edilizia penitenziaria.

il parere è contrario. Esso è volto a modificare la disciplina in materia di destinazione

finalizzato ad affrontare il problema reale dell'utilizzo delle macchine agricole per finalità diverse da quelle strettamente riconducibili alle attività agricole, rischiando di mettere in discussione tutto il sistema delle immatricolazioni e di prestarsi anche a qualche utilizzo abusivo, naturalmente non voluto dai proponenti ma che oggettivamente si porrebbe ove la norma venisse approvata. Quindi, il parere è contrario.

ha motivato la sua opposizione, con la quale concordo, facendo riferimento alle isole minori, mentre nel testo in esame leggo - a meno che non ci sia un'*errata corrige* di cui non sono in possesso - isole maggiori.

Anzi, è un argomento su cui ha richiamato la nostra attenzione - se non sbaglio - nella seduta della settimana scorsa il senatore Storace, quando si è soffermato in particolare sul problema degli stanziamenti per elicotteri a favore dei trasferimenti con le isole minori.

Prescindendo da questi chiarimenti di carattere più che altro terminologico e pur preannunciando voto contrario, vorrei sottolineare che i collegamenti fra la Sardegna e il continente rappresentano risalente ma ancora attuale, e credo che bene abbiano fatto i presentatori dell'emendamento a presentarlo alla nostra attenzione. Ricordo - il mio ricordo risale, però, ad almeno a 40 anni fa - una presa di posizione dell'allora presidente della Repubblica Segni, il quale si pronunciava già su questo tema e sosteneva una tesi forse oggi non più attuale, ossia la necessità e l'opportunità di estendere i traghetti delle Ferrovie dello Stato alla Sardegna che all'epoca non esistevano. Credo che a quel tempo non fosse nemmeno operativo il collegamento con Golfo Aranci. il rimedio non è forse quello indicato dall'allora presidente della Repubblica Segni, ma certamente il problema rimane: resta il fatto che l'emendamento qui proposto, al di là delle difficoltà di copertura, pone pone problematiche di armonia con il resto dell'articolo, che ha tutta una sua coerenza. Questo, che è presentato come comma aggiuntivo, in realtà è un vero e proprio articolo aggiuntivo che tratta temi diversi da quelli trattati dall'articolo.

brevemente per aggiungere la mia firma all'emendamento 34.3, presentato dal collega Fantola ed altri, non solo perché non è non è riservato esclusivamente alla Sardegna e parla di isole maggiori, ma perché pone il tema delle Autostrade del mare, tante volte enfatizzato dal Governo come strumento alternativo ad un Piano di infrastrutture e di collegamenti che, per esempio, riguardano anche la Regione Sicilia. Il *lapsus* freudiano del relatore sulle isole minori mi serve per confutare la tesi proposta qualche minuto fa dal collega secondo il quale questo disegno di legge finanziaria conterrebbe misure adeguate per le isole minori:

Presidente, chiedo un po' di attenzione, perché l'argomento è molto delicato ed il collega della maggioranza l'ha fatto presente nell'assoluto disinteresse - come mi è sembrato - del Governo e del relatore, che ha commesso un errore madornale: ha parlato di isole minori.

FI).* State portando avanti, cioè, un ingiustizia madornale: invece di parlare di continuità territoriale, mettendo nelle stesse condizioni tutto il trasporto, escludete l'unica Regione che purtroppo non ha alternative. Mi rivolgo allora alle persone serie, come il collega della maggioranza, affinché correggano il Governo ed il relatore, che - forse perché è molto stanco? - ha parlato di isole minori, che non c'entrano assolutamente niente con la Sicilia e la Sardegna. Mi rivolgo soprattutto ai parlamentari sardi: cosa farete? Voterete contro questo emendamento, l'unico che, per la prima volta, dà qualcosa anche alla Sardegna (non solo alla Sardegna, ma anche alla Sardegna)? Non è possibile, infatti, che i nostri autotrasportatori

che per trasportare i prodotti ed i manufatti devono pagare il doppio. Ecco perché che su questo tema vi richiamo ad un atto di onestà: 77 milioni di euro all'anno, per tre anni; zero alla Sardegna, pochissimo alla Sicilia. Se votate contro, vi dovrete vergognare!

di lavoro, di fare un riferimento non appropriato ad una tipologia di isole. Chiedo scusa, ma il parere rimane contrario per evidenti problemi di copertura a finanziaria.

Presidente, poiché il testo dell'emendamento ha un contenuto molto dettagliato con molti riferimenti normativi, come ho già detto al senatore Battaglia,

in Commissione dell'emendamento 35.0.3 che riguarda la problematica dei progetti di finanza, cioè la ritenuta necessità di reintrodurre il diritto di prelazione per il promotore, elemento questo che costituirebbe secondo i proponenti un elemento di forte attrattività per questo tipo di realizzazioni di opere pubbliche. Credo che se il senatore Grillo presentasse un ordine del giorno in tal senso se ne potrebbe valutare l'accoglibilità, considerando che l'esigenza che lui pone è condivisa, intervento normativo adesso, a pochi mesi dalla modifica del codice dei contratti pubblici, non è invece ancora maturo.

tentativo razionale e impegnativo per il Governo di organizzare sul piano pluriennale una manovra di infrastrutturazione nelle aree meridionali, attraverso una dotazione finanziaria congrua e rispettando le previsioni di una delibera del CIPE, che, facendosi carico dell'arretratezza e del *deficit* infrastrutturale, elemento straordinariamente penalizzante per tutto il sistema sociale ed economico dell'area meridionale che tutti a parole considerano l'unico fattore attraverso il cui sviluppo possa innestarsi una vera crescita strutturale dell'economia del Paese, sia sul terreno della domanda interna che dell'occupazione, che sul piano di una capacità di competizione dell'intero sistema economico nazionale. A queste ripetute affermazioni di principio non consegue però alcuna attività concreta. Quella delibera del CIPE che ho richiamato, per quanto posso considerarla simbolica e manifesto, rappresenta l'espressione di una volontà politica importante, quella di ancorare i finanziamenti per le infrastrutture ad una percentuale

la necessità di ripensarla e di modificarla in termini normativi, fissando in modo congruo le risorse e imponendo questa scelta. che non vorrei ascrivere semplicemente alla volontà della classe politica e della rappresentanza meridionale, ma che dovrebbe diventare patrimonio politico dell'intero Paese, se c'è davvero il convincimento che esiste una condizione di *deficit*, di debolezza infrastrutturale ed economica del Mezzogiorno che è questione nazionale. Questa mi sembra una buona occasione per incominciare ad invertire la tendenza.

Siete gli autori, i fautori del mantenimento dello Stato centralista e noi ci troviamo in finanziaria con il cappello in mano a chiedere l'elemosina per portare a termine delle

*(FI)*. Presidente, faccio appello ai riformisti del centro-sinistra. Questo emendamento non comporta dei costi, ma riproduce una condizione che si è consolidata nel 2003, 2004, 2005 e 2006. Al Nord si sono fatte importanti opere pubbliche con il coinvolgimento di capitali privati. In questo modo si è alleggerito il bilancio dello Stato, che quindi ha avuto più risorse per investire al Sud. Eliminare il diritto di prelazione significa,

realizzare opere pubbliche. Nelle città del Nord i parcheggi, i termovalorizzatori, le piscine, gli impianti sportivi, le carceri, gli ospedali ormai si fanno con la tecnica del *project financing*. a parer mio, il ministro Di Pietro, per incultura o per una svista grossolana che ha compiuto il 31 luglio, ha avallato una decisione che ha azzerato questa condizione, questo principio e questa norma.

Sull'emendamento 36.7, senatore Castelli, esprimo parere favorevole: la possibilità di introdurre la destinazione in via prioritaria delle risorse per l'edilizia penitenziaria agli edifici esistenti mi sembra una soluzione di buon senso.

intervengo per esprimere poche parole di apprezzamento per questo articolo, che si occupa di interventi strutturali e di ammodernamento tecnologico in diversi settori, da quello scolastico a quello penitenziario. Desidero appuntare l'attenzione, però, sul settore sanitario. L'articolo 36 passerà anche con alcuni emendamenti che sono stati approvati in Commissione bilancio. In primo luogo, sono stati previsti 3 miliardi in più per gli interventi strutturali in campo

per occuparsi di quelle persone che vengono dimesse dall'ospedale, per assisterle quindi dopo la fase acuta della malattia. Accanto a questo, però, gli emendamenti che sono stati approvati in Commissione bilancio vanno ad interessare parte di questi 3 miliardi che sono stati previsti dal Ministero della salute e voluti in modo particolare dal ministro Turco e destinati a due momenti particolari della vita delle persone: il momento iniziale e il momento finale.

circa 40 patologie per le quali è possibile avere una cura a disposizione e siamo in grado di consentire a questi bambini di crescere in una condizione di quasi normalità.

per le cure palliative e per le situazioni di coma. Credo che queste scelte dimostrano la volontà del Governo di porre attenzione anche a quei temi eticamente sensibili

dove da questa mattina sono scesi in assemblea i lavoratori che non hanno una percezione del loro futuro. Abbiamo l'obbligo l'obbligo di dare una mano a quei lavoratori e di programmare anche il futuro di Malpensa. Guardate che se la gallina smette di mangiare in Padania, se noi non la facciamo mangiare, finisce anche di fare le uova d'oro

e su quello che versa come tasse. Datecene indietro una piccola parte per fare quelle infrastrutture delle quali siamo carenti da

perché è corretto che l'Aula sappia che questa passerà alla storia del Parlamento come la finanziaria che ha introdotto i maggiori privilegi a favore delle imprese cinematografiche. Va bene organizzare le cose in maniera tale che costoro paghino meno tasse, va bene che costoro abbiano più contributi, ma adesso volere imporre che i film italiani debbano andare in prima serata, che le televisioni private siano obbligate a collocare nel loro palinsesto nelle prime ore della serata i film perché prodotti dai cineasti italiani mi sembra veramente assurdo. Torniamo indietro di parecchi anni, in una logica tutta assistenzialista di uno Stato che pretende di governare cosa devono fare le televisioni private, tutte, quelle grandi quelle grandi e quelle piccole. Mi pare una vera e propria esagerazione, per cui un poco di buonsenso dovrebbe consentire a quest'Aula di correggere accogliendo l'emendamento che mi sono permesso di proporre. *(Applausi

intervenite in modo estremamente punitivo nei confronti delle televisioni che hanno l'accesso condizionato, dove cioè l'utente compra e guarda quello che vuole quando vuole: è un obbrobrio.

nei confronti di queste categorie. Se volete tener fede agli impegni assunti da un anno e mezzo nei confronti di tutti, sottoscrivetelo e votatelo, perché è un atto di coscienza che voi stessi vi dovete riconoscere visto che ci siamo battuti per queste categorie.

dei malati affetti da altre patologie indicate nel testo dell'emendamento. Tuttavia, i colleghi ricorderanno che quando approvammo l'emendamento al decreto,

di un emendamento identico a quello di cui stiamo discutendo oggi, insieme ad altri colleghi ha determinato di presentare un ordine del giorno, votato all'unanimità in Commissione bilancio. In esso si invita il Governo ad affrontare, nel prosieguo della sessione di bilancio, questo tema

nei prossimi passaggi della legge finanziaria. Quindi, invito i colleghi dell'opposizione, oltre che a considerare che la maggioranza condivide questo

Confermo quanto ebbi modo di dire nel corso della discussione sul decreto, Confermo quanto ebbi modo di dire nel corso della discussione sul decreto, e cioè che

Il Governo ha iniziato ad affrontare il problema con lo stanziamento nel decreto ed intende affrontarlo in modo strutturale attraverso i cosiddetti programmi pluriennali

avevo fatto riferimento al corso della legge finanziaria che inizia al Senato e prosegue alla Camera. Quindi, confermo l'impegno ad affrontarlo alla Camera

Presidente, colleghi, questo emendamento è la conseguenza di una altra votazione che abbiamo fatto, sulla quale il Parlamento ha preso una posizione Contrario il relatore, contraria la ministra Turco, quest'Aula ha stabilito che chi ha avuto danni irreversibili alla persona ed è in causa contro le aziende sanitarie di questo Paese,

al punto che la ministra aveva chiesto al primo firmatario Marino di ritirare l'emendamento perché pensava che la copertura non fosse sufficiente. Era pure vero,

In Aula, però, è stato detto che ci avrebbe pensato la finanziaria, perché il decreto stabiliva solo 150 milioni per il 2007, che sono insufficienti. Abbiamo fatto una promessa vana. Abbiamo preso in giro tantissime persone *(Applausi non portiamo avanti la nostra posizione, nel senso di riconoscere quel diritto, e non si vuole trovare in finanziaria i soldi sufficienti, siamo la burla del Paese.

del Senato. Al di là degli schieramenti e dei riti di parte, esistono impegni ben precisi, ossia dei risarcimenti che non possono più essere compensati con gli inviti rivolti al Governo. rivolti al Governo. Stiamo parlando di persone che non hanno più tempo. Probabilmente questa maggioranza avrà una nuova finanziaria sulla quale investire in termini di promesse elettorali. Fuori da questa Aula ci sono persone che hanno diritto ad essere risarcite. L'appello è rivolto a tutti quei senatori che hanno a cuore un impegno preciso assunto con quanti sono stati danneggiati a nome e per conto di una cattiva sanità che purtroppo ancora esiste nel Signor Presidente, non vorrei inserire toni ulteriormente polemici nei confronti del Ministro, perché parliamo di una questione maledettamente seria.

all'emendamento che quest'Aula approvò all'unanimità. Qui voglio dare atto del coraggio e della presa di posizione responsabile del presidente Marino in quella serata. Votammo all'unanimità. Il relatore ci dice che adesso non è il tempo: quand'è il tempo, signor relatore, di varare un provvedimento a favore di malati che attendono che lo Stato dia loro una mano? Questo è il tempo: nel decreto abbiamo approvato misure per l'anno in corso; qui si sta dicendo che, per gli anni a venire, dobbiamo aiutare queste persone. Ho colto positivamente il fatto che il ministro Turco abbia chiesto la parola, prima: mi sarei aspettato almeno un atto, un gesto con cui dicesse che, pur non essendo in grado di impegnare per dieci anni il bilancio dello Stato, almeno andava bene stanziare 180 milioni per il prossimo anno, per dare la possibilità a questi malati di vedere la luce. E invece nemmeno questo! Ecco perché spero che questo emendamento sia approvato, perché non è giusto incontrare questi malati ogni giorno e contraddirli in quello successivo.

ramo del Parlamento ha manifestato grande sensibilità - anche se nei limiti delle possibilità di allora, temporalmente circoscritte - ci sta molto a cuore.

bisogna trovare coperture adeguate, altrimenti poi sollevate la polemica sul fatto che sforiamo i parametri, e così via. Mi domando se non sia possibile accantonare questa norma, in modo che il relatore ed il Governo possano possano individuare, almeno per il prossimo anno, una copertura adeguata al fine di venire incontro ad un problema che effettivamente è drammatico; alcuni di noi lo sanno anche per esperienza indiretta, ma vicina; comunque ci è a tutti noto.

Presidente, se la risposta è quella dell'accantonamento, non posso che dichiararmi soddisfatta della soluzione. Quello che però mi disturba nella discussione svolta qui questa sera sono certi accenti abbastanza esagerati, perché all'interno della Commissione abbiamo svolto un lavoro serissimo, anche di ampliamento delle categorie interessate al problema. Quindi, la volontà di trovare una soluzione c'è e il Ministro l'ha sottolineata.

Però, in chiusura di seduta - anche perché lei vorrà apprezzare le circostanze - vorrei segnalare ai colleghi una necessità. Sul fatto che occorre risolvere problemi così importanti e seri è da anni che discutiamo e non solo in finanziaria; che si preveda una spesa di 1.800 milioni per i prossimi dieci anni, mi sembra possa risolvere un annoso problema. Però, Presidente, tutti i colleghi dovrebbero anche imparare, oltre a prevedere le misure sulle quali bisogna fare le spese, anche a fare uno sforzo sul reperimento delle risorse finanziarie. Mettere una copertura che taglia ancora una volta nel settore oggettivamente è una non copertura. Allora è troppo facile anche per l'opposizione e qualche volta per la maggioranza

Le finanziarie hanno tanti difetti perché c'è questa pessima abitudine di volere una cosa e non dire da dove prendere i soldi. Mi auguro che tutti insieme, maggioranza e opposizione, facciamo uno sforzo per reperire le risorse necessarie perché scaricare tutto sul Ministro è una comodità che non ci possiamo permettere.